recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

Signora Presidente, onorevoli senatori, intendo ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti ed, evidentemente, anche coloro che hanno prestato attenzione alla discussione generale. Tra coloro che sono intervenuti, un accenno merita il senatore Gentile che, molto efficacemente, ha fissato secondo cui il provvedimento non va nella direzione di migliorare le condizioni economiche delle banche, quanto di impegnare le banche, all'occorrenza con il sostegno del Governo,

direttamente al sistema produttivo. Ella ha perfettamente ragione e poiché la fiducia, come tutti i sentimenti, come l'amore, non si possono fissare per legge, evidentemente la sua sollecitazione, come quella degli altri colleghi che vanno in questa direzione con il loro pensiero, può servire per esercitare quella *moral suasion* necessaria affibché chi ha orecchie intenda e chi deve operare operi per assecondare il risultato che la filosofia di questo provvedimento intende conseguire. La senatrice Spadoni Urbani ha ripetuto, grosso modo, le stesse perplessità sicché, ancora una volta, chi leggerà gli atti di questa discussione (sono fiducioso che gli uffici studi degli enti competenti, prima fra tutti la Banca d'Italia, non mancheranno di farlo) saprà quali sono le aspettative che il Parlamento italiano assegna a questo benefico provvedimento governativo. Il senatore Firrarello poi ha ricordato il grande sacrificio compiuto dal Mezzogiorno d'Italia quando ha subito la settentrionalizzazione del sistema bancario. Caro senatore, esprimo comprensione ed affetto. Auguriamoci che nel tempo l'intero sistema bancario, ma anche le autorità di Governo che di volta in volta saranno chiamate alla funzione, si ricordino - quando sarà scritta la storia economica del Mezzogiorno d'Italia - che l'evento più grave è stato

opportunamente ha esternato l'opinione, a volte diffusa, che la dirigenza di qualche banca debba prestare più attenzione alle politiche dei dividendi e ai compensi per i *manager*.

che una soluzione per traslare i benefici effetti di questo provvedimento al sistema produttivo può essere quella di dare incentivi al personale. Ebbene, noi siamo convinti che all'ufficio fidi delle banche non manchino le domande di richiesta di concessione di credito. Può mancare, piuttosto, una sorta di audacia che nei momenti di crisi viene meno in coloro che debbono erogare il credito e che noi auspichiamo riaffiori, considerato che il Governo ha fatto il suo dovere per intero mettendo, per dirlo con una frase molto pittoresca, il suo portafoglio sui conti dei depositanti e quindi sui debiti delle banche. il senatore Vaccari ha rappresentato l'apprezzamento per il provvedimento governativo, mentre il senatore Morando, che ci ha deliziati con una conversazione di politica economica, ha suggerito qualcosa che, a mio avviso, rappresentanti del Governo, merita di essere tenuta in conto: la possibilità che parte dei fondi rivenienti da questo provvedimento possa essere applicata per potenziare i consorzi fidi. Se è vero che per la via dei consorzi fidi è più facile dare serenità e audacia alle banche che devono concedere i finanziamenti, è evidente che se una porzione di queste risorse la si utilizza per questo apparato, che noi da non molto tempo abbiamo voluto ridisegnare con un provvedimento legislativo pregevole e che ha dato i suoi più egregi risultati, certamente è un fatto oltremodo positivo. La senatrice Germontani ha ribadito il principio della finalità di questo provvedimento, che va nella direzione della tutela del risparmio. Per concludere, rappresentanti del Governo e amici, agli atti di questo Parlamento rimarranno queste istanze e queste aspettative, tutte pregevoli e condivisibili, che vanno nell'unica direzione di apprezzare il provvedimento e di sperare che i suoi effetti possano spiegare benefica azione a favore del sistema produttivo. Io sono convinto

Non è casuale che il sistema bancario italiano fosse stato tutto riordinato utilizzando questo strumento, di cui abbiamo imparato l'espressione tanto tempo fa, che a volte ci ha dato dispiacere quando ha determinato la settentrionalizzazione del sistema bancario, ma evidentemente questa tattica di persuasione, la *moral suasion*, è tanto efficace e tanto valida che ha determinato una ristrutturazione che mai la storia economica aveva potuto registrare.

dibattito che ha ampliato il tema, contenuto nel decreto‑legge, su una serie di decisioni di politica bancaria e finanziaria. Noi abbiamo Noi abbiamo detto, nella presentazione del provvedimento, nella discussione alla Camera e poi in quella in Commissione al Senato, che il provvedimento aveva una finalità molto particolare: porre fine a quell'effetto panico che si era generato nel Paese a fronte dell'esplosione della bolla finanziaria che si è verificata a metà settembre negli Stati Uniti e in Europa e che, verso la fine di settembre, in Italia aveva avuto il momento di maggiore forza. In quei giorni c'era il rischio - era successo in Inghilterra, stava accadendo anche nel nostro Paese - che ci fosse una caccia ai depositi da parte dei risparmiatori italiani e che il ritiro dei depositi bancari nel Paese provocasse un effetto *default* complessivo sul sistema finanziario nazionale che avrebbe provocato la crisi del sistema. Il provvedimento è nato a fronte di questa emergenza, tanto è vero che esso contiene che esso contiene due norme: la garanzia dello Stato a fronte dei depositi fatti dai cittadini italiani nei confronti delle banche italiane fino alla cifra già garantita dall'assicurazione interbancaria, che però in quei giorni non era più considerata una garanzia sufficiente da parte della maggioranza dei cittadini italiani, e la possibilità dello Stato di intervenire nel capitale delle banche, nel caso in cui si andasse verso una situazione Il provvedimento contiene anche una garanzia dello Stato a fronte del mercato interbancario per cercare di far ripartire il mercato stesso. In quei giorni c'era anche un effetto panico non solo dei risparmiatori nei confronti delle banche, ma anche dei singoli banchieri, che tendenzialmente non si scambiavano più il denaro l'un l'altro. Questa era la filosofia contenuta nel provvedimento, che abbiamo cercato di mantenere. Da quei giorni la crisi Da quei giorni la crisi finanziaria ha avuto un impatto negativo anche sui mercati finanziari complessivamente e sull'economia reale. Sapete che si è ridotta un po' la concessione di credito delle banche specialmente alle piccole e medie imprese; il Governo, a fronte del sistema di concessione di credito italiano,

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta. La Commissione osserva che il testo fonda la propria straordinaria connotazione, sia per quanto riguarda i profili di copertura che per quanto concerne l'attuazione della spesa attraverso provvedimenti di natura amministrativa - difficilmente inquadrabile nei normali parametri di giudizio della legge di contabilità dello Stato - sulla eccezionalità della congiuntura internazionale che ha registrato anche in altri Paesi europei interventi del medesimo segno».

ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.5, 3.0.7 e 5.0.4 (limitatamente alla lettera *e)*). Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4 e 4.0.2. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte».

Signora Presidente, sinceramente non capisco la ragione di un pronunciamento avverso. Questo ordine del giorno non fa altro che dare suggerimenti ed indicazioni circa la necessità che, per esempio, per quanto attiene agli studi di settore e all'applicazione degli interventi di carattere fiscale nei confronti delle piccole e medie imprese e libero-professionali, si usi una misura che tenga conto dell'andamento della situazione economica. Tra l'altro, un indirizzo che anche nel decreto-legge n. 185, assunto dal Governo, è esplicitato come dichiarazione di intenti. Qui si va nella direzione di dare qualche indicazione più precisa

Ieri il senatore Morando è intervenuto in discussione e credo sia stato apprezzato da tutti il senso della sua riflessione circa la necessità e l'importanza di costruire dei meccanismi che diano fiato e rafforzino il ruolo dei confidi.

visto che l'ordine del giorno va nella direzione di allentare quelle che possono essere considerate delle maglie troppo strette da parte del sistema bancario nei confronti

rispetto ad un tema che in questo caso non riguarda i risparmiatori singoli, ma può coinvolgere quelle amministrazioni pubbliche che, magari non per responsabilità loro, come è avvenuto anche a tanti singoli sottoscrittori,

a tempo indefinito per effetto di una situazione che si spera possa essere recuperata e corretta. Si tratta quindi di individuare una qualche soluzione tecnica temporanea che sterilizzi almeno in parte l'effetto negativo dell'andamento del ciclo economico di

PD)*. Colleghi, vi chiedo cortesemente di non votare per chi è assente.

Onorevoli colleghi, avverto che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono inammissibili, per estraneità alla materia trattata dal decreto-legge in esame, i seguenti emendamenti: 1.5, 1.13, 1.14, 4.11, 4.0.3, 5.0.5 e 5.0.6. Analoga decisione è stata assunta anche nel corso della discussione presso la Camera dei deputati. La Presidenza consente tuttavia ai presentatori di illustrare le ragioni che li avevano indotti a sottoscrivere gli emendamenti dichiarati inammissibili.

tra i depositi raccolti e gli impieghi verso lo Stato per acquistare valori mobiliari azionari di società quotate, senza diritto di voto nelle assemblee ordinarie per quattro anni dalla data d'acquisto.

per offrire misure di stabilità e fiducia ai risparmiatori sul sistema bancario.

mutuatari di abitazioni di residenza che siano temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o di comproprietari. In sostanza, si chiede di mostrare attenzione ad un profilo di socialità

(una metodologia che serve per rinforzare e ricapitalizzare le banche, ma non può essere utilizzata in questa fase di intervento pre-insolvenza, che necessita invece di un intervento di capitale),

per informare l'Aula che in Commissione finanze era stato raggiunto un accordo per trasformare alcuni emendamenti in ordini del giorno.

si dà una cambiale in bianco, una fideiussione *omnibus* alle banche che continuano ad incamerare *stock* *options*. cifra di 26.000-27.000 euro al giorno per uno dei primi banchieri e di oltre 450.000 azioni di una delle più grandi banche

**Il Senato non approva.**

la sollecitazione dei colleghi ha indotto il Governo ed anche il relatore a riconsiderare l'opinione su alcuni ordini del giorno. In particolare,

insiste sempre sulle stesse questioni. In effetti, tutti gli emendamenti che abbiamo presentato a questo articolo vanno nella direzione di rafforzare i fondi a sostegno della possibilità di consentire l'accesso al credito o di facilitare, in un momento di congiuntura negativa, l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, particolarmente per

Ricordo a me stesso, all' Assemblea, al relatore e al rappresentante del Governo che tale formulazione era già contenuta in una disposizione emanata dal Governo Prodi

Trovo particolarmente incongruo, singolare, che il nuovo Governo, in particolare il ministro Tremonti, abbia ritenuto di cassare questa tipologia di potenziali utilizzatori e beneficiari dello strumento, avendone stravolto in qualche modo anche le caratteristiche, sia ampliando la platea dei potenziali beneficiari sia arrogando a se stesso la possibilità

Mi sembra una procedura molto censurabile e ritengo grave il fatto che si sia unilateralmente deciso di mortificare e danneggiare una categoria di risparmiatori.

L'attuale Governo si trincera spesso dietro le decisioni attribuite al Governo Prodi (penso alla questione dell'IVA sulle televisioni,

precluso il minimo spiraglio di una speranza di recuperare una parte del danno subìto. Immagino siano diverse le situazioni di questo genere in Italia; io ne conosco una riferita alla mia Regione. Sinceramente ritengo che quei cittadini, quei risparmiatori guardassero con un po' di speranza alla possibilità

una punta di maliziosa cattiveria e di astioso compiacimento, che mi sembra l'esercizio di un potere interpretato in modo piuttosto

ci troviamo di fronte a titoli che erano stati garantiti con il massimo dell'affidabilità, ossia la tripla A,

i titoli della Lehman Brothers ed altri 47 titoli "tossici" erano consigliati con il massimo dell'affidabilità.

una breve illustrazione di questo emendamento, che riguarda sempre

affrontiamo riguardano le lacrime e il sangue della gente, dei richiedenti il credito, che sono vessati da un sistema bancario che dovrebbe riformarsi e che non può solo

favorevole sull'ordine del giorno

l'emendamento 5.3. Stiamo in questo periodo prendendo decisioni che servono ad attrezzare gli organi di Governo per poter tempestivamente intervenire e fronteggiare situazioni di difficoltà, anzi, in qualche caso le misure tardano a venire rispetto a quella che sarebbe l'intensità della crisi, come abbiamo detto nel dibattito e diremo nella dichiarazione di voto

L'emendamento 5.3 tende a stabilire, pur rispettando l'esigenza di decidere in fretta, un percorso di monitoraggio e di interlocuzione più rafforzato, con un coinvolgimento maggiore

delicati, con decisioni e decretazioni che possono avere implicazioni particolarmente rilevanti.

problema che abbiamo a lungo discusso anche con il presidente Baldassarri e con il presidente Azzollini, ossia alla mediazione creditizia.

per difendere quel sistema famiglia che la Lega Nord ma spero tutti quanti consideriamo come il perno della nostra società. ricordare a me stesso e rileggere le parole del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, il 15 luglio scorso, pertanto poco tempo fa.

per portare ordine e sicurezza nelle attività svolte dagli intermediari finanziari non bancari, e dalla moltitudine incontrollabile di mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. aggiungeva che i requisiti per l'accesso al mercato da parte di questi operatori e gli strumenti di controllo a disposizione delle autorità non sono in grado di assicurare adeguati livelli di qualità del servizio e non consentono un efficace presidio contro i rischi di illegalità e di contiguità con le attività criminose. Il numero spropositato degli iscritti, oltre 1.200 intermediari e circa 160.000 agenti e mediatori, conferisce al fenomeno dimensioni preoccupanti (sono sempre parole del governatore Draghi). Aggiungeva che l'allarme sociale destato dalle operazioni di Polizia, che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazione della normativa antiriciclaggio e di frodi, richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico. Penso che queste siano parole assolutamente pesanti e mi rivolgo al Governo perché si tenga in considerazione di porre mano a questa normativa che è assolutamente stringente

gli ordini del giorno G101 e G102. Accoglie come raccomandazione

Volevo solo segnalare questa anomalia e vi prego di notare che lo faccio dopo l'accadimento, per non mettere in difficoltà né la Presidenza, né la volontà della persona; ma credo che le regole vadano rispettate, anche perché

questa venga cancellata semplicemente con un ordine del giorno che - come si sa - è come un sigaro: non si rifiuta a nessuno.

è stata cassata tutta la procedura della tracciabilità dei pagamenti, vorrei chiedere se all'interno del Governo vi sia il segno di un ripensamento che, ovviamente, saluterei con particolare entusiasmo. Mi sembrava giusto richiamarlo all'attenzione dell'Aula: sarebbe molto opportuno andare in questa direzione e non solo per quanto attiene ai versamenti agli agenti assicurativi.